Sospendo pertanto la seduta fino alla conclusione dei suoi lavori. *(La seduta, sospesa

sarà discussa la mozione Bonino ed altri sull'istituzione di una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Il calendario prevede lo svolgimento del sindacato ispettivo nelle giornate di mercoledì 11, martedì 17 e giovedì 26 luglio e lo svolgimento del *question time* giovedì 12 e giovedì 26, alle ore 15, con trasmissione diretta televisiva. Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 19 luglio, alle ore 14,30, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Nella settimana dal 17 al 19 luglio sarà discusso, ove concluso dalla Commissione, il decreto-legge sulla fatturazione elettronica delle cessioni delle cessioni di carburante. Previo accordo con la Camera dei deputati, nella giornata di mercoledì 18 luglio, alle ore 9,30, sarà indetta la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione della RAI. Sempre nella giornata di mercoledì 18 luglio - che è il mio compleanno - *(Applausi)*, alle ore 12, avranno luogo le votazioni a scrutinio segreto,

Nella settimana dal 24 al 26 luglio sarà esaminato il decreto-legge recante interventi per il tribunale di Bari, ove approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto riguarda le sedute uniche di mercoledì 18 e mercoledì 25 luglio, i lavori dell'Assemblea saranno tendenzialmente sospesi tra le ore 13 e le ore 16,30 per consentire il lavoro delle Commissioni.

i Gruppi che non abbiano già provveduto facciano pervenire le designazioni dei propri rappresentanti nella Commissione di vigilanza RAI, nel Copasir, nonché nella Giunta delle elezioni e delle immunità

Entro lunedì 23 luglio dovranno pervenire le designazioni dei Gruppi nelle delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali; entro lunedì 30 luglio, le designazioni concernenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali e le altre Commissioni bicamerali previste dalle leggi vigenti, che si rinnovano a inizio legislatura.

Si tratta di un'interrogazione che riguarda l'ENAV e le scelte dell'ultimo piano industriale, che stanno agitando da tempo i suoi dipendenti, ma anche i passeggeri. Se, da una parte, è stato scongiurato lo sciopero di tutti i controllori di voli di ventiquattr'ore del prossimo 5 luglio, c'è da essere ancora seriamente preoccupati per il rinvio al 20 luglio dello stesso sciopero: rischiamo di dar vita a un venerdì nero al contrario del traffico aereo, considerando gli effetti devastanti per l'industria delle vacanze di uno sciopero all'inizio di un fine settimana di metà luglio. Le organizzazioni sindacali di ENAV riferiscono che, da quando questa società ha fatto il suo ingresso in Borsa, appare con sempre maggiore evidenza la propensione a tagliare e accorpare servizi, in ragione di una tutela dei conti e degli utili da parte dell'azienda, di quella che è la reale missione di ENAV, ossia provvedere alla sicurezza nei cieli. A triste conferma di questa inclinazione, lo scorso 1° luglio si è registrata una giornata orribile per il traffico aereo italiano, dovuta a un'avaria ai sistemi di controllo del centro *radar* di Roma: proprio il centro designato dal piano industriale di ENAV quale unico - e sottolineo unico - *radar* per il Centro e il Sud Italia. una scelta che va commentata e valutata con la notizia che, proprio grazie alla ridondanza *radar* messa in atto dal centro di controllo di Brindisi, che si vuole chiudere in via sperimentale a brevissimo giro, si è riusciti ad accompagnare i voli in corso e a limitare i ritardi e i disagi.

quali sono gli intendimenti riguardo alle scelte di gestione che ENAV sta compiendo, la cui portata è di rilevante importanza per la sicurezza dei nostri cieli e dei cittadini.

Signor Presidente, l'intervento mi si rende indispensabile oggi a seguito delle incredibili dichiarazioni dell'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari,

Va bene per l'assessore Montanari e per la sindaca Raggi trasformare la città in una discarica a cielo aperto, quale è oggi Roma - è sotto gli occhi di tutti - per la gioia di topi e cinghiali, ma non deve essere chiuso - secondo loro - il ciclo dei rifiuti. È chiaro che tutta l'area metropolitana di Roma e la Regione Lazio sono pronte e devono fare la loro parte per dare una mano a risolvere i problemi; altra cosa è pensare che l'area metropolitana di Roma, i Comuni della Provincia di Roma e i Comuni del Lazio vengano trasformati in discariche per i rifiuti di Roma.

di tantissime capitali europee, non riesca a risolvere il problema del ciclo dei rifiuti, portando i rifiuti all'estero o in altre Regioni e chiamando sempre alla solidarietà altre situazioni, con un costo

il segretario della Lega e vice *premier* Matteo Salvini a venire in quest'Aula a chiarire la gestione dei rimborsi elettorali, che pure oggi la stampa nazionale attribuisce

tutto ciò. Pensiamo che le dichiarazioni del segretario della Lega e vice *premier* Salvini dovrebbero rappresentare un sufficiente incentivo alla Presidenza per invitare il Ministro a chiarire i fatti in Aula. Che cosa ha detto? Ha detto che le risorse e il tempo speso dalla magistratura per queste indagini sono buttati via e che i soldi dei rimborsi sono già stati spesi. Non solo: oggi,

il Ministro debba venire in Parlamento a chiarire. Sono affermazioni rese da una persona che ha giurato sulla Costituzione per diventare Ministro c'è veramente qualcosa di fatto male, perché la separazione dei compiti e delle competenze tra la magistratura e il Governo è un principio sancito dalla nostra Costituzione. Signor Presidente, mi sembra che si stia prendendo una china

si fa tutto fuori dal Parlamento e per lo stretto necessario si viene qui, anche se questo stretto necessario è veramente poca cosa, visti i ritmi di lavoro delle ultime settimane. Ebbene, per noi la questione Lega-Salvini vice*premier* è una questione di sostanza e come tale va

anni e anni di malagestione ci hanno lasciato in eredità situazioni catastrofiche e disastrose, a partire da quella dei precari dei centri per l'impiego. Si tratta di una piaga che ha dell'assurdo, perché le stesse persone che dovrebbero aiutare gli altri nella ricerca di un lavoro vivono la preoccupazione di non averne uno stabile. Ma non è tutto perché, in questo sventurato passato, alla malagestione si è unita anche la «malalegislazione»: dal dicembre 2014 si è assistito a un vero e proprio smantellamento del personale, a eccezione di L'Aquila. Poi è arrivato il decreto Madia, che non ha fatto altro che generare altre disparità. Ad oggi i precari abruzzesi dei centri per l'impiego scontano dei requisiti di stabilizzazione diretta fortemente pregiudizievoli e criteri di implementazione del personale che non hanno considerato adeguatamente le graduatorie già esistenti, nonostante esse siano valide, perché prorogate sin dal 2014 dalle varie leggi di stabilità. Il risultato è che nelle tre province di Chieti, Teramo e Pescara manca attualmente il personale e di conseguenza non sono assicurati i livelli essenziali delle prestazioni: una delle mille contraddizioni che, e instancabile attività del nostro ministro Di Maio, siamo pronti a spazzare via. La segnalazione che mi arriva è stata fatta da quei lavoratori e da quelle famiglie in difficoltà e non cadrà nel vuoto, Presidente, perché il vento è cambiato. Ribadisco con fierezza quello che ripetiamo da anni e che è scritto nero su bianco nel nostro contratto di Governo: i centri per l'impiego saranno potenziati su tutto il territorio nazionale, incrementandone la presenza, l'efficienza e la qualità dei servizi. Allo stesso tempo saranno adeguati anche i livelli formativi del personale operante. Concludo, Presidente: la strada è tracciata e noi ci impegneremo al massimo affinché tutti lavoratori, anche quelli che operano nei centri per l'impiego, non continuino a vedere calpestati i propri diritti. *(Applausi

è di pochi giorni fa la notizia che, con il ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea, il Parlamento europeo vorrebbe ridurre il numero dei deputati da 751 a 705 in vista delle elezioni del 2019. Contestualmente vi è la proposta, in seno alla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, di una di una nuova redistribuzione dei seggi che assegnerebbe all'Italia tre posti in più. Questa notizia, a noi valdostani in particolare, non è passata inosservata. l'unica Regione italiana ad avere la quasi certezza di non essere mai rappresentata a Bruxelles o a Strasburgo nel Parlamento europeo, in quanto inserita in un grande collegio del Nord-Ovest, che, dal punto di vista numerico, ci obbliga, ogni volta che ci sono le elezioni europee, ad apparentarci, con risultati quindi totalmente inefficaci e inutili. motivo per cui negli ultimi giorni, anzi proprio ieri, ho ripresentato un disegno di legge, con alcuni aggiornamenti, che propone l'obiettivo di creare una circoscrizione specifica per la Valle d'Aosta in occasione delle elezioni europee, proprio come fecero i Padri costituenti quando previdero, nello Statuto di autonomia valdostana, di creare i collegi uninominali per le elezioni politiche. Quindi, vista l'importanza che tutti noi conosciamo per siffatto argomento, chiedo fin d'ora il sostegno di tutte le forze politiche presenti in questa Assemblea, affinché, con un atto di autentica democrazia, anche la più piccola Regione del nostro Paese, che rappresenta un popolo che abita le terre più alte d'Europa, e quindi con necessità e problematiche del tutto particolari, possa avere la dignità di una sua rappresentanza nel Parlamento europeo per contribuire - noi lo sosteniamo da sempre, da convinti federalisti - a far nascere una vera Europa dei popoli.

Signor Presidente, desidero riportare in tempo reale lo studio che è stato eseguito in queste ore sulla disastrosa alluvione, che ha interessato

dunque all'attenzione questo aspetto, che deve essere affrontato, perché il cambiamento climatico sta rendendo molto meno efficaci le opere idrauliche che abbiamo realizzato. Si tratta quindi di un problema che dobbiamo mettere in conto, per